nessuno mette in discussione la necessità di riformare, ristrutturare e razionalizzare la rete consolare italiana nel mondo.

Questi dubbi sono tali che hanno portato la Commissione affari esteri ad accogliere un'altra proposta che abbiamo fatto, che è quella di un'indagine conoscitiva sul funzionamento della rete consolare italiana nel mondo e del Ministero degli affari esteri. Colgo l'occasione per chiarire - perché ne abbiamo parlato solo in Commissione - ed insistere sulla parola: noi abbiamo chiesto, ed è in atto, un'indagine conoscitiva, e non punitiva. Deve infatti essere chiaro l'obiettivo di questa indagine: vogliamo acquisire gli elementi necessari per fare il nostro ruolo di rappresentanza in questo Parlamento e contribuire a definire un nuovo impianto, una nuova rete consolare e un nuovo concetto dei servizi, con il Governo. Questo è l'obiettivo. Questa indagine è iniziata da pochi giorni, ed è anche nata dalla presentazione di una riforma del Ministero degli affari esteri che - credo di non offendere nessuno nel dirlo

si chiede questo periodo di fermo per permettere al Parlamento di svolgere la sua normale funzione di conoscere e proporre (poi ognuno assumerà le proprie responsabilità nelle decisioni finali),

e siamo coscienti che bisognerà trasformare questa rete). Tutto ciò però creerà dei problemi notevoli all'amministrazione e al funzionamento di questi uffici, in un periodo con scadenze elettorali importanti, come quelle dei *referendum* o delle prossime elezioni politiche. Il termine puntava così

proporrei una riformulazione che preveda un termine dell'ordine di 12 mesi per la moratoria, oppure, in alternativa, la conclusione dell'indagine conoscitiva

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, prendo la parola, nonostante non partecipi all'attività della Commissione affari perché sento la responsabilità, di fronte a questa mozione, di quanto è scritto all'articolo 67 della Costituzione, e cioè che noi qui in Parlamento rappresentiamo, tutti insieme, la Nazione senza vincolo di mandato: rappresentiamo quindi i cittadini elettori che vivono in Italia e gli elettori italiani che vivono fuori dall'Italia, nel mondo. Sappiamo che i nostri colleghi eletti nei collegi all'estero sono in prima fila sul tema che oggi discutiamo, ma è ma è bene che sappiano che non sono soli, che tutti noi siamo con loro. I consolati italiani, ma anche gli istituti italiani di cultura all'estero, sono strumenti fondamentali per far vivere l'Italia tra gli italiani che sono nel mondo, ma anche per far vivere l'Italia nel mondo.

(dobbiamo sapere che in questi mesi è cresciuta nelle università di tutto il mondo la domanda di studio della lingua italiana), della sua musica. Noi dobbiamo pensare a un circuito unico in Italia e all'estero, a una grande sinergia. Mi viene in mente l'intuizione di Giuseppe Dossetti di alcuni decenni fa: una politica estera che è sempre anche politica interna. Questo fatto lo si è visto nelle celebrazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia, un evento globale che ha varcato i confini del nostro Paese e che ha fatto sentire ancor più forti negli italiani che vivono all'estero le radici dei luoghi di provenienza, dei focolari lontani da cui si è partiti insieme e anche l'appartenenza a una sola comunità nazionale. La rete consolare, dunque, anche grazie alla passione e alla competenza dei suoi operatori, è un servizio indispensabile per gli italiani residenti all'estero, di prima e seconda generazione, che hanno portato in ogni parte del mondo l'umanità dell'Italia, il lavoro, la cultura.

Questi italiani si sono mescolati al resto del mondo, ed è nato così questo nostro tempo degli ultimi due secoli, fatto dall'intreccio di culture diverse. diverse. Di fronte a queste riflessioni, dobbiamo semplicemente guardare al piano di ristrutturazione di questa rete. Valutiamolo bene: lo facciamo per risparmiare risorse? Non credo: anche il sottosegretario Mantica lo ha riconosciuto. In difesa dei consolati minacciati di chiusura da questa riorganizzazione si muovono le città in cui essi hanno sede. Ho avuto l'opportunità di vedere di recente a Lille, in Francia, i COMITES di tutta la regione

Si è mobilitata la città di Lille e il suo sindaco, una donna di grande valore come Martine Aubry, ha scritto una lettera al ministro Frattini: il consolato, ha scritto, è essenziale non solo per gli italiani ma per tutta la popolazione, per l'economia della zona e per il dialogo interculturale nel cuore dell'Europa, perché Lille è esattamente lì. In questi giorni i COMITES di Francia, ricordando i 150 anni dell'Italia unita, hanno scritto una lettera aperta al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato e al Governo: la loro è una supplica accorata.

si faccia un quadro chiaro delle sedi; si migliorino le condizioni operative e comunicative; si dia forza all'Italia nel mondo. Questa è oggi la nostra responsabilità verso gli italiani che vivono fuori dall'Italia, verso l'Italia stessa, verso il mondo. Sostenere la rete con la visione del futuro senza rinunciare al valore degli italiani elettori all'estero, non vorrei che anche iniziative improvvide fossero la spia che è in gioco ciò che abbiamo conquistato: con lo smantellamento dei consolati, anche la presenza dei cittadini elettori italiani nelle sedi fuori dall'Italia. Se, come credo, condividiamo il senso dell'espressione «Italia nel mondo», allora è opportuno che ci fermiamo a riflettere per trovare insieme le soluzioni migliori,

Signor Presidente, signor sottosegretario Mantica, egregi colleghi, intervengo anche a nome dei colleghi eletti nella circoscrizione Estero per segnalare che andiamo fieri all'estero della gestione fatta della crisi economico-finanziaria da parte del nostro Paese, che ci ha permesso di uscire da quel terribile acronimo dei cosiddetti Paesi PIGS, sostituendo la «I» d'Italia con la «I» di Irlanda. Quindi, condividiamo in linea di massima l'attenzione che bisogna portare alla ristrutturazione della spesa dello Stato. Però, nello specifico di questa amministrazione, non possiamo non notare che i tagli lineari sono stati suddivisi dall'amministrazione del Ministero degli affari esteri in modo ineguale a sfavore degli interessi degli italiani all'estero. sia corretto: innanzitutto perché gli italiani all'estero sono coloro che hanno contribuito di meno alle cause principali del nostro dissesto finanziario, nel senso che non hanno certo contribuito alla creazione del debito pubblico; luogo, perché si tratta di una comunità in crescita. Gli italiani all'estero sono di più che in passato perché continuiamo ad emigrare e, nel momento in cui continuiamo a farlo, i tagli alla struttura diplomatico-consolare sono tanto più gravi. pensiamo di chiudere un consolato che interessa 60.000 italiani per riunirlo a quello di Ginevra, dove risiedono 40.000 italiani; a Manchester si chiude un consolato dove risiedono 30.000 italiani; ad Amburgo 15.000 italiani; a Lille - che è stata citata, ma ci sono le autorità locali di tante circoscrizioni consolari che hanno scritto a noi e alle nostre autorità, non solo Lille: quasi tutte, in realtà - 30.000 persone; a Liegi 53.000 persone insistono sul consolato che si andrebbe a chiudere; a Mons 35.000. Nell'ambito di tali ragionamenti, quindi dell'ortodossia economico-finanziaria di cui noi anche all'estero andiamo fieri, portata avanti dal Governo, ma anche nell'ottica delle necessità specifiche

per contribuire all'analisi delle iniziative di razionalizzazione degli uffici diplomatici e consolari» e ad «avviare (...) un confronto con le Commissioni parlamentari competenti per una valutazione strategica del ruolo della rete Quella del senatore Pedica impegna il Governo «ad approfondire il progetto di riordino della rete degli uffici all'estero», nonché alla «rivisitazione dei compiti e delle funzioni delle numerose istituzioni che oggi rappresentano ed operano in favore dei cittadini italiani all'estero» tenendo presenti: «l'importanza strategica di taluni uffici (...)», il «ruolo delle nuove tecnologie nel processo di ammodernamento delle procedure amministrative» ed «il necessario e costruttivo confronto con il Parlamento».

tutti i consolati italiani saranno dotati di un nuovo sistema informativo per la gestione degli sportelli. Per chi è esperto di consolati, ciò significa che gli sportelli consolari non hanno più

nei consolati nei quali è stato installato (cito Berlino e Berna), un miglioramento del servizio che rendiamo ai nostri utenti da questo punto di vista. Preciserò poi qualcosa in merito. I parlamentari sanno perfettamente che, una volta realizzato questo impianto (torno a sottolineare che, al 31 dicembre 2011, tutti i consolati italiani avranno il sistema dovrebbe essere approntato (un primo esempio è stato già illustrato alle Commissioni a Bruxelles) quello che noi chiamiamo, in analogia con un servizio che credo molti senatori utilizzino, l'*home banking*. Si tratta della possibilità

mantenendo inalterati i servizi e investendo in informatica (è evidente che non si tratta solo di *software*, ma anche di *hardware* che deve essere distribuito). In questo quadro, credo che possa essere valutata - o almeno, così il Governo la valuta - in maniera diversa

i 600.000 visti del consolato di Mosca non riguardano gli italiani nel mondo. La competenza del consolato di Abu Dhabi, il quale svolge attività sostanzialmente commerciali,

modo, mi rendo conto che si è focalizzata l'attenzione sui consolati che servono alle comunità italiane nel mondo, e possa interessare poco al Senato che il Ministero degli affari esteri sta aprendo una sede di ambasciata ad Ashgabat ed una a Giuba.

o erano di poco interesse per noi, come Ashgabat, la capitale del Turkmenistan, che pare abbia qualche giacimento di gas e petrolio che in questo momento hanno un certo interesse strategico. Se ragioniamo in una visione più ampia e complessa, forse riusciamo a trovare un'intesa su questo tema.

vorrei un giorno aprire un dibattito in questa sede e capire che cosa voglia dire essere emigrato italiano in un Paese della Comunità europea, dove esiste la Patria europea, o dove lavoriamo per costruire il senso di cittadinanza europea.

questa è una battaglia di tipo politico ed amministrativo, che rende il mondo dell'Europa, e dei servizi che in essa dobbiamo rendere, non direttamente paragonabile a quello - ad esempio - dell'Australia, del Sud Africa o dell'America latina. Torno a ripetere che la chiusura attuale dei consolati programmati riguarda solo l'Europa, e non gli italiani nel mondo. Vengo ad un'altra osservazione, di carattere dialettico.

Altra osservazione, a cui tengo molto, perché ci sono delle occasioni di carattere politico nelle quali non si può usare l'espressione «l'abbiamo persa».

Per legge abbiamo presentato in Parlamento la ristrutturazione e aperto un dibattito, che è durato meno di quattro ore.

Le occasioni perse non è che poi si ritorcono qui su altri argomenti, perché è chiaro che in quella sede la ristrutturazione della rete poteva avere un altro significato, in quanto si inseriva nella ristrutturazione del Ministero. Ma anche questo lo capisco.

I numeri hanno un significato, un senso. Ragioniamo su quelli e sulla valutazione dei costi e dei servizi. Perché scrivere: «Si produrrà così lo spostamento dalle sedi chiuse alle nuove sedi di competenza di centinaia di migliaia di pratiche»?

data alla realizzazione di quello che chiamiamo il progetto del servizio consolare a distanza, che ho cercato di spiegare prima, paragonabile all'*home banking*. Questo, per rimarcare e sottolineare

Se gli atti notarili all'estero li facciamo pagare un quinto di quanto li fa pagare il Comune di Lille, è probabile che i servizi al consolato italiano aumentino moltissimo. Mi domando se sia corretto che facciamo un'operazione di *dumping* di percezione consolare in giro per il mondo avendo poi decine di migliaia di persone che vengono nei nostri uffici a chiedere i servizi.

cui sono condizionati sino alla data del 31 marzo 2012 i provvedimenti di revisione della rete consolare non ancora formalmente deliberati dal consiglio di amministrazione

di aumentare l'efficienza dei servizi dei consolati attraverso l'uso degli strumenti che la tecnologia ci mette oggi a disposizione.

al fine di costruire un progetto condiviso di profonda riforma della rete e dei servizi consolari italiani nel mondo e di rispettare pienamente i diritti democratici degli italiani residenti all'estero». In pratica, tale nella sua formulazione così come presentata dai firmatari della mozione, con l'inserimento classico dei limiti imposti dal bilancio e dalla conseguente

a elaborare sue proposte o sue valutazioni - e il raggiungimento di un obiettivo di carattere tecnologico o di efficienza dei servizi. Se la riformulazione proposta dal Governo fosse accettata dai firmatari, la mozione si intende ovviamente

che questi sono più utili per l'Italia in altri Paesi, ai quali accennava prima il Sottosegretario, credo siamo tutti d'accordo. Utilizzo un'immagine molto semplice, Presidente: in Europa non abbiamo bisogno della diplomazia del Ferrero Rocher,

è un'indagine conoscitiva. Se l'abbiamo chiesta è perché forse il dialogo che c'è stato con l'Amministrazione degli esteri nella presentazione del piano di riforme del Ministero non ha convinto la Commissione, che ha accolto tale richiesta

dobbiamo andare avanti con il piano di ristrutturazione. Accetto la riformulazione che propone il Governo, a dimostrazione che questa mozione non ha niente di strumentale, ma è l'espressione di una volontà di lavoro congiunto.

il funzionamento dello sportello informatico, che può funzionare: ci dobbiamo solo rendere conto di chi può accedere a un servizio informatico, visto che i nostri emigrati non hanno un'età

rappresenti e difenda gli interessi del proprio Paese all'estero offrendo servizi a tutela delle comunità italiane nel mondo. Non dimentichiamo che l'organizzazione e la presentazione degli uffici di rappresentanza all'estero costituisce in molti casi, insieme agli istituti italiani di cultura, il biglietto da visita del nostro Paese, condizionando sensibilmente la promozione delle politiche del turismo verso l'Italia. Il piano di ristrutturazione della rete consolare, prevedendo la chiusura di alcune importanti sedi, tra cui Lille, Losanna, Liegi, Amburgo, Filadelfia e Detroit, peggiorerà la funzionalità di una rete consolare già in difficoltà. Sul tema sono stati espressi critiche e dubbi in tutte le sedi, comprese quelle parlamentari, da parte degli addetti ai lavori, e soprattutto da parte dei rappresentanti italiani all'estero, all'estero, anche per portare avanti questa mozione, presentata e condivisa da tutti noi. La 3a Commissione permanente del Senato ha deliberato all'unanimità la realizzazione di un'indagine conoscitiva che ha come obiettivo quello di conoscere l'effettiva situazione dell'organizzazione dei servizi e della rete diplomatico-consolare italiana all'estero. si vuole impegnare il Governo a promuovere nell'immediato uno specifico provvedimento di moratoria che differisca per un termine di 12 mesi il piano di ristrutturazione presentato dal Ministero degli affari esteri e a congelare la rete consolare nella sua attuale situazione, nonché a tenere conto dell'esito dell'indagine conoscitiva della 3a Commissione permanente del Senato sulle strutture del Ministero, al fine di costruire un progetto condiviso di profonda riforma della rete e dei servizi consolari italiani nel mondo e di rispettare pienamente i diritti democratici degli italiani residenti all'estero. L'unico punto che il Gruppo Italia dei Valori non condivideva riguardava la lunga moratoria di 30 mesi prevista nella prima versione della mozione, perché rischiava di configurare unicamente una scusa per il Governo di essere inoperativo.

«sino alla data del 31 marzo 2012 i provvedimenti di revisione della rete consolare non ancora formalmente deliberati dal consiglio d'amministrazione Questa non è una moratoria, perché ciò significa che le delibere assunte su Losanna, Liegi ed altri consolati vanno avanti lo stesso. Non credo che lo spirito di collaborazione si possa chiedere fino a questo punto.

nuova finestra"). Saluto gli studenti dell'Istituto paritario «Maddalena di Canossa», di Brescia, che sono in visita al Senato,

sulla struttura centrale e periferica del nostro Ministero degli affari esteri, anche se dobbiamo procedere a tappe, a causa della molteplicità dei problemi che

ad una ristrutturazione importante di tutto quanto il Ministero degli affari esteri è e fa, in Italia e all'estero. Ieri abbiamo parlato della rappresentanza degli italiani all'estero; è in corso una riflessione sulla partecipazione sindacale dei funzionari assunti a tempo determinato nelle istituzioni all'estero, secondo le leggi dei Paesi di loro residenza; oggi continuiamo una riflessione sulla ristrutturazione della rete degli uffici all'estero, studiando le tre componenti che fanno parte di tale ristrutturazione: le risorse umane, la diffusione territoriale ed i servizi prestati. dunque non solo della chiusura di consolati e ambasciate o di immobili, ma anche - ed ecco l'elemento nuovo - di una ristrutturazione delle sedi materiali, con il relativo riassetto della distribuzione delle risorse umane nel territorio, che avviene grazie all'introduzione di un progetto di informatizzazione della prestazione dei servizi consolari.

Questo progetto di prestazione di servizi a distanza per via informatica è idoneo ad eliminare molti disagi per gli utenti e anche a mettere una soluzione alla molteplicità di uffici e di servizi che noi abbiamo.

ha lasciato insoddisfatti una parte di coloro i quali sono intervenuti e, soprattutto, non ha completamente soddisfatto il primo proponente della mozione. Comprendiamo che non si tratta

la decisione finale su questo provvedimento di un termine molto breve. La prossima settimana potremmo infatti riprendere e, mi auguro, concludere positivamente e con l'accordo di tutti

Presidente, credo che sia necessario un rinvio, per permettere al Governo di portare

vuol dire però che noi dobbiamo ascoltare cosa ci vengono a dire sistematicamente le amministrazioni più che

Mantengo inoltre con grande convinzione, malgrado le difficoltà, questa disponibilità al dialogo, purché ci mettiamo d'accordo

Quando ho scritto che è già stato comunicato "l'atto di chiusura ed è stato ottenuto l'assenso dalle autorità di accreditamento", significa che di questo si è già parlato con la Repubblica federale tedesca,

C'è stata anche un'interruzione nei colloqui con la Repubblica federale tedesca, di cui è perfettamente informata tutta la comunità nazionale, essendo perfino intervenuto il sindacato dei contrattisti a termine nella Repubblica federale tedesca.